la seduta antimeridiana di giovedì 13 novembre è stata tolta senza l'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 12 novembre. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 13 novembre, bisogna approvare il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 12 novembre. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Invito ora il senatore Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 13 novembre.

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 dicembre.

Una volta concluso tale provvedimento, riprenderà - sempre nella giornata di oggi - la discussione generale del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, possibilmente fino alla sua conclusione. A tal fine l'orario di chiusura della seduta pomeridiana è previsto per le ore 22. Diversamente, la discussione generale potrà concludersi domani mattina. Non appena pervenuto il parere della Commissione bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni previste dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sulla conformità alle regole di copertura del disegno di legge finanziaria, trasmesso dalla Camera dei deputati. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni presenteranno, entro le ore 16 di giovedì 27 novembre, i propri rapporti alla 5a Commissione permanente che concluderà 1'esame in sede referente entro sabato 6 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 10 di lunedì 8 dicembre. La discussione in Aula inizierà nella seduta antimeridiana di martedì 9 dicembre. Il calendario della trattazione in Assemblea e la relativa ripartizione dei tempi saranno successivamente definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. Nel corso di questa settimana sarà discusso il decreto-legge in materia di lavori pubblici, autotrasporto e agricoltura. Il calendario della settimana è poi integrato - acquisita 1'unanimità tra i Gruppi ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento - con l'esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente. Nel pomeriggio di giovedì 20 novembre si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata sulle infrastrutture nel Mezzogiorno, con particolare riguardo al ponte sullo stretto di Messina. La prossima settimana, dal 25 al 28 novembre, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge in materia di lavori pubblici, saranno discussi gli altri decreti-legge presentati in prima lettura al Senato in materia di rilancio del settore agroalimentare e di università, per i quali si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Saranno inoltre poste all'ordine del giorno relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di insindacabilità. Nella settimana successiva alla prossima, dal 2 al 5 dicembre, saranno esaminati i decreti-legge approvati e trasmessi dalla Camera dei deputati concernenti crisi dei mercati finanziari internazionali, disagio abitativo e emergenza rifiuti in Campania. Il calendario delle prossime settimane potrà essere integrato con l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Si fa presente che, tenuto conto dei numerosi e impegnativi provvedimenti pendenti, il calendario di questa e delle prossime due settimane prevede sedute con votazioni dal martedì mattina al venerdì pomeriggio e pertanto non è prevista sospensione dei lavori dell'Assemblea in concomitanza con la sessione di bilancio. Peraltro, gli orari delle sedute sono stati impostati in modo tale da lasciare congrui spazi per i lavori delle Commissioni impegnate nell'esame dei decreti-legge, dei documenti finanziari e dei provvedimenti collegati, con particolare riguardo al federalismo fiscale. Tali spazi potranno essere eventualmente rivisti in relazione al concreto andamento dei lavori. Ricordo infine che in apertura della seduta pomeridiana di domani sarà commemorata la figura di Alma Cappiello, già componente della nostra Assemblea, a due anni dalla sua scomparsa.

che il Gruppo dell'Italia dei Valori non è rappresentato all'interno del Consiglio di Presidenza. Noi riteniamo che questo sia un fatto assolutamente grave per un Gruppo come il nostro, composto da 14 senatori

con riferimento al calendario che avete approvato - dove risulterà anche la nostra assenza, quindi la nostra non approvazione, come abbiamo specificato - vorremmo chiederle alcune modifiche rispetto ai lavori

Fratini risponde: «Mica sono stupido: l'avrebbe fatto anche lei! Stiamo comprando l'Alitalia senza soldi e fra tre anni guadagneremo 300 milioni. La maggior parte di noi ha messo solo la firma, rischiamo solo in caso di bancarotta, di nostro non rischiamo nulla».

dall'opposizione (dunque dal Partito Democratico e dall'Italia dei Valori), il disegno di legge sulla sicurezza è stato in qualche modo bloccato nel suo *iter* di approvazione qui in Senato.

vorrei invece chiedere ai colleghi Capigruppo di fare tutti un passo indietro, prendendo atto anche della posizione dell'Italia dei Valori, che ha chiesto di non partecipare, anzi, ci riferisce che non parteciperà più alle prossime Conferenze dei Capigruppo, perché in disaccordo

ulteriormente compresso e limitato i tempi della nostra discussione in Commissione. La maggioranza ha ritirato gli emendamenti, che poi riproporrà in Aula, ma noi non sappiamo quale sia l'orientamento del Governo su tali proposte e lo apprenderemo in questa sede. Noi stessi abbiamo dovuto

circa l'integrazione del Consiglio di Presidenza, devo far rilevare al senatore Bricolo che non si tratta di una richiesta di posti

Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal collega Zanda e credo che il tema vada sgomberato da questioni che hanno un'importanza e un rilievo politico e istituzionale di gran lunga superiori.

Devo dire però, senza vena polemica, ma rivolgendo un invito ai colleghi dell'Italia dei Valori, che non credo sia opportuno non partecipare alla Conferenza dei Capigruppo per il mancato posto di Segretario di Presidenza, visto che siamo tutti d'accordo nell'affrontare e risolvere la questione. che è minima rispetto ad un calendario dei lavori - che abbiamo approvato ed il cui voto a favore riconfermiamo in quest'Aula - che dà la precedenza assoluta ai temi economici e finanziari, che sono la vera priorità di questo Paese. in particolar modo, alla legge finanziaria e ai disegni di legge collegati alla finanziaria, su cui abbiamo opinioni diverse. Ma poiché ci troviamo in una fase di crisi profonda del sistema economico e produttivo anche italiano, riteniamo che la prima priorità per le famiglie italiane sia quella di ottenere da noi risposte concrete, efficaci ed immediate, soprattutto in sede di legge finanziaria, a tali problemi. Per tale ragione abbiamo sostenuto e sosteniamo questo calendario dei lavori e credo che tutti dovremmo recuperare il senso della realtà e della concretezza della situazione che il Paese sta affrontando in questi mesi.

oltre 160 senatori hanno fatto proprio un appello al Governo italiano per cancellare dalla lista delle organizzazioni terroristiche il gruppo dei Mujaheddin del popolo iraniano. All'interno di quel documento vi era anche una richiesta di particolare attenzione relativamente ad un campo profughi nella città di Ashraf, al confine tra Iraq e Iran. Da stasera sarò in viaggio nell'ambito di una delegazione non ufficiale, ma militante, che si recherà a Ashraf. Tale comprende anche il vice sindaco di Cuneo, militanti e dirigenti del Partito radicale nonviolento e di "Nessuno tocchi Caino". Questo perché, come tutti saprete, nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Governo iracheno secondo il quale il controllo delle zone urbane alle forze nazionali. Esistono enormi problemi di sicurezza per 3.500 persone e la nostra presenza in quei luoghi vuole, in qualche modo, rispondere fattivamente alle richieste avanzateci dai Mujahedin del popolo nelle settimane scorse, sperando però che in futuro una delegazione ufficiale

per evitare un intervento armato in Iraq, preferendo l'opzione, che poi fu da più parti boicottata, di mandare Saddam Hussein in esilio. Ebbene, se allora quell'atto di coraggio, sollecitato da un'iniziativa di Marco Pannella, fosse stato preso in considerazione pienamente e politicamente, oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Spero che questo sia, se non altro, il mio penultimo intervento in Aula. Esso vuole valere in parte anche come testamento biologico. *(Commenti dai banchi conoscono le mie opinioni in merito, essendo uno dei firmatari delle proposte di legge che verranno discusse, ma essendo anche ottimista spero di poter contribuire all'adozione di quel progetto.

riguardante una scelta della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, che ha restituito i beni immobili che erano in custodia di molti usurati agli usurai.

dopo che sono stati condannati gli usurai, attraverso l'interpretazione della sezione misure di prevenzione del cosiddetto pacchetto sicurezza, questi beni vengano restituiti agli usurai. Erano beni di proprietà degli usurati, che gli usurati avevano in custodia!

che dà la stura ad un meccanismo di restituzione di beni a moltissimi usurai nel territorio, criminalizzando di fatto le vittime di usura.

E questaesigenza di rappresentatività è tanto più avvertita da noi in quanto abbiamo una considerazione "maggioritaria" della dialettica e della dinamica all'interno del Senato.

ciò. D'altra parte, abbiamo notato che all'interno del Regolamento i margini affinché ciò fosse consentito erano estremamente ristretti, anzi inesistenti.

far presente, sotto il profilo della pura razionalità, che dal punto di vista istituzionale la situazione oggi non sarebbe stata differente se fosse stato eletto un membro dell'Italia dei Valori e non un membro dell'altro Gruppo.

ostruzionistico nei fatti non riconosca quello che, invece, la maggioranza autonomamente ha riconosciuto. Quindi, nel ribadire in Aula l'impegno affinché le esigenze di rappresentatività siano soddisfatte, invito i colleghi del Gruppo Italia dei Valori a rivedere il loro atteggiamento perché renderebbe più facile e più fluido lo svolgimento del lavoro in Senato. Signor Presidente, abbiamo ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti i Capigruppo. Vorrei essere molto chiaro: il tema - e l'ho specificato poc'anzi - non è

Tutto il resto lo abbiamo già notificato e credo che debba restare agli atti. Signor Presidente, è soltanto la notifica di quello che sta accadendo: noi chiediamo una modifica del calendario dei lavori che voi avete approvato.

che, all'inizio della seduta, si dia la parola effettivamente su temi inerenti l'ordine dei lavori e non altro. Questa mattina ho concesso facoltà di intervento a tutti i colleghi anche su altri argomenti perché non erano resi edotti, ovviamente, della decisione della Conferenza dei Capigruppo e quindi

temi posti, abbiamo ritenuto tutti, con la massima condivisione, che all'inizio della seduta gli interventi sull'ordine dei lavori siano attinenti al tema reale dell'andamento dei lavori. Detto questo, oggi ho ricevuto una lettera del collega Belisario che anticipava la mancata presenza alla riunione dei Capigruppo,

Il tema lo conosciamo, è stato ampiamente spiegato nella nota, e ha sempre toccato la sensibilità di questa Presidenza: la garanzia di una presenza parlamentare di tutti i Gruppi negli organi interni di funzionamento del Senato. Oggi - lo ricordava il senatore Quagliariello - abbiamo ampliato la Giunta per il Regolamento, consentendo la presenza dei rappresentanti dei Gruppi ancora non presenti, quali il senatore Belisario, il senatore Pistorio, il senatore D'Alia, proprio volendo dare il senso della volontà della Presidenza, che è quello di garantire a ciascun Gruppo la rappresentanza negli elementi decisionali interni al Senato che non siano l'Aula e le Commissioni, e che poi attengono da un lato all'interpretazione del Regolamento, dall'altro lato (mi riferisco al Consiglio di Presidenza) al funzionamento dell'apparato Senato. Quindi è stato fatto un passo che non è altro che l'attuazione del pensiero della Presidenza,

che ha avuto la possibilità di competere alle ultime elezioni, ha avuto consensi, si è costituito nella propria totale identità, che quindi esiste e naturalmente reclama il diritto di una rappresentanza nel Consiglio di Presidenza, che non ha potuto avere attraverso il voto della settimana scorsa. Ho anche invitato i Gruppi, in sede di Giunta per il Regolamento, a farsi carico di eventuali iniziative. Apprezzo gli interventi dei senatori Zanda e D'Alia, cioè di esponenti dell'opposizione, che hanno condiviso questa esigenza. Posso assicurare il senatore Giambrone che

Pertanto (anche se non c'è il presidente Belisario lo dico al senatore Giambrone, che in questo momento sta fungendo da vice), mi permetto di rivolgere un forte invito

una lettera. PRESIDENTE. Non esistono precedenti e non è rituale un dissenso preventivo su quello che si sta discutendo. Sarebbe stata sufficiente - mi permetto di aggiungere

Prendo atto che sia il Gruppo dell'Italia dei Valori sia quello del Partito Democratico non si sono detti disponibili ad una scelta di questo tipo e che restano dunque nella posizione di bloccare di fatto

Caro senatore Zanda, dal momento che prima si è riferito anche al mio intervento, voi avevate fatto un accordo con il Gruppo Italia dei Valori, voi avete tradito quell'accordo visto che la settimana scorsa, quando avete votato, 40 voti (40 voti!) del suo Gruppo sono stato dirottati sul candidato del Gruppo Misto e non su quello dell'Italia dei Valori. È inutile, quindi, che adesso lei rivendichi

il disegno di legge sulla sicurezza non andrà avanti e che questo Senato continuerà a discutere dei problemi delle poltrone dell'opposizione, che evidentemente gli stanno più a cuore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in titolo reca la conversione del decreto-legge 25 settembre disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Tale decreto-legge deve essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il 25 novembre

alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 fino alla piena operatività della nuova concessione e, comunque, non oltre il 1° luglio 2009. La suddetta previsione rappresenta l'ultima di una serie di proroghe inaugurate dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). con un bando del 29 giugno 2007, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha messo a gara la procedura di selezione per l'affidamento in concessione per nove anni dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Alla gara hanno partecipato SISAL, Lottomatica e SNAI. Con un successivo decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della SISAL S.p.A. A tal fine, la SISAL ha effettuato, nella scorsa primavera, una ristrutturazione finanziaria della società. Come riportato nella relazione al disegno di legge di conversione, Enalotto. La gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all'individuazione di un nuovo concessionario (SISAL S.p.A.) che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle delle sue attribuzioni, perché si deve attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari che garantiscano l'idoneità della nuova organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il decreto-legge è stato integrato con l'aggiunta degli articoli 1-*bis* e 1-*ter*. L'articolo 1-*bis* (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse) interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero agli altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica

È prevista una riduzione dell'importo da corrispondere, pari al 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta, qualora le concessioni vengano aggiudicate a soggetti già titolari

il 2003, la possibilità di effettuare scommesse all'interno degli ippodromi anche su corse tenute in altri campi viene estesa alle scommesse a quota fissa (mentre oggi ciò è consentito per le sole scommesse a totalizzatore); inoltre, tale possibilità non viene più limitata ai giorni di svolgimento delle gare, sopprimendo quindi ogni vincolo temporale. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, un fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio e la raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Con un apposito decreto, si prevede che una parte delle risorse di tale fondo venga destinata, in primo luogo, all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e, in secondo luogo, anche alle progressive esigenze finanziarie relative all'attività istituzionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata nei bilanci dello Stato. Viene stabilito inoltre, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'incremento del prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) dal vigente 12 per cento al 12,70 per cento delle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del suddetto incremento rispetto alle entrate relative all'anno 2008 sono assegnate all'UNIRE, per essere interamente destinate all'incremento del montepremi. Si dispone, inoltre, l'assegnazione all'UNIRE di un contributo, per il solo anno 2008, di 25 milioni di euro, al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali del medesimo ente. Per far fronte a tale onere si prevede la corrispondente riduzione del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali. Si stabilisce inoltre la destinazione all'incremento del montepremi delle eventuali ulteriori maggiori entrate, rilevate annualmente dall'AAMS, derivanti dall'attuazione del presente articolo 1-*bis*. Per effetto di una modifica apportata alla legge finanziaria per il 2005, si introduce anche il divieto di scommettere su manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. Gli eventi su cui non sarà più possibile scommettere sono quelli organizzati dalle associazioni

L'articolo 1-*ter* (Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito) rimette ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina relativa alla sperimentazione di apparecchi elettronici per il gioco lecito collegati in rete. Si tratta degli apparecchi facenti parte della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. il medesimo decreto ministeriale sono dettate, altresì, le norme per la sperimentazione e la raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi. Il medesimo articolo 1-*ter* reca l'interpretazione autentica di una norma della legge finanziaria per il 2006, al fine di determinare con esattezza il compenso erogato ai concessionari della rete telematica a titolo di corrispettivo dell'ammodernamento degli apparecchi da gioco e della raccolta dei dati di funzionamento. Si segnala, da ultimo, che la Commissione finanze della Camera aveva introdotto - con l'approvazione dell'emendamento governativo 1.02 - un ulteriore articolo in materia di esercizio e raccolta a distanza (*on line*) dei giochi in Italia, in cui si prevedeva l'emanazione di appositi regolamenti atti a disciplinare *ex novo* o ad adeguare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza di una serie di giochi analiticamente indicati nel dettato normativo. Tale articolo, però, è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'Aula della Camera. Il Governo si è riproposto di presentare, in tempi ravvicinati, un apposito disegno di legge sul tema, tenuto conto dell'avvio nei confronti dell'Italia di due procedure di infrazione comunitaria relative alle proprie modalità di gestione del gioco a distanza. *(Applausi

Informo il Senato che questa mattina avrà luogo solo la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fontana. Ne ha facoltà.

Governo, ancora una volta ci troviamo ad affrontare in quest'Aula un disegno di legge di conversione di un decreto-legge del Governo, prassi - quella dell'uso della decretazione d'urgenza - che sta assumendo in modo sempre più consolidato e preoccupante la caratteristica di normalità e ordinarietà di questi primi mesi di legislatura. Ancora una volta, si parte con un decreto che ha una determinata finalità (in questo caso, assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi); questo viene firmato dal Presidente della Repubblica e successivamente, nel corso dell'esame in Commissione, il Governo presenta emendamenti che stravolgono il testo iniziale, inserisce articoli aggiuntivi di consistente rilievo, che modificano sostanzialmente il contenuto del decreto e che meriterebbero ben altra attenzione e maggiore cautela. Ancora una volta, quindi, uno schiaffo al ruolo del Parlamento, al nostro ruolo, messi come siamo nella condizione di non riuscire a svolgere compiutamente il nostro lavoro e ad affrontare con la dovuta serietà l'esame dei provvedimenti. Serietà tanto più necessaria quanto più siamo chiamati ad esaminare materie oggettivamente complesse e delicate, estremamente importanti dal punto di vista economico e che producono un effetto sociale di massima rilevanza. Il decreto-legge interviene infatti in un settore - quello dei giochi e delle scommesse - che ha un giro d'affari di 42 miliardi di euro di fatturato all'anno (quasi il 3 per che ha fatto registrare un incremento pari al 19,7 per cento nel 2007 rispetto all'anno precedente e del 169 per cento dal 2003 al 2007. 42 miliardi di euro all'anno, circa 720 euro giocati ogni anno da ogni cittadino italiano, compresi i neonati. E se a questo aggiungiamo i dati dell'indagine della Guardia di finanza, che da sola ha accertato fatturati illeciti di circa 43 miliardi di euro, è evidente la portata di ciò di cui stiamo parlando. Si tratta, inoltre, di un settore che ha subito e sta subendo trasformazioni radicali e in rapidissima evoluzione, attraverso la massiccia introduzione delle tecnologie telematiche, che stanno determinando un vero e proprio boom di giochi e scommesse *on line* dove, tra l'altro, pullulano siti di scommesse non autorizzati. Non possiamo non rilevare in questa sede che il profilo del giocatore tipo in ambito *web* fa registrare un notevole incremento del numero dì giovani tra i 18 e i 26 anni. Si tratta, altresì, di un settore per la cui regolamentazione lo Stato non può non tenere conto dei risvolti etici estremamente delicati che esso implica, se solo pensiamo alle dimensioni che il fenomeno della dipendenza da gioco e scommesse ha ormai assunto nel nostro Paese, una vera e propria patologia, un'emergenza sociale che coinvolge non solo il giocatore ma anche tutta la sua famiglia e, in particolare, i soggetti più deboli. Ebbene, crediamo che proprio la complessità di una materia come questa, i diversi piani di lettura e i diversi interessi in campo su cui dobbiamo cercare di trovare un equilibrio, le implicazioni di ordine economico, occupazionale, sociale ed etico, la coerenza con il quadro normativo europeo, insomma, tutta questa complessità avrebbe meritato un percorso decisamente diverso da quello che ci viene proposto dal Governo. Sono convinta che unanimemente riconosciamo l'esigenza di stabilire un preciso assetto normativo in materia, di evitare il perpetuarsi di ricorrenti modifiche alla disciplina e di produrre un quadro legislativo stabile, necessario tanto per l'amministrazione quanto per gli operatori, volto ad assicurare una tutela adeguata ai consumatori, utile a contrastare il pericoloso fenomeno del gioco irregolare o illegale e della sua contiguità con la criminalità organizzata. In sostanza, riteniamo occorra intervenire in modo organico sulla materia e, del resto, anche il sottosegretario Giorgetti in questi giorni ha annunciato in Commissione la presentazione di un disegno di legge organico sulla materia. Ma è proprio per questo che non è minimamente giustificabile l'inserimento nel decreto di ulteriori modifiche, in alcuni punti anche poco chiare e certamente improvvisate. Sul testo originario del decreto legge, che conteneva un'unica disposizione riguardante una proroga della concessione per il gioco dell'Enalotto al fine di non interromperne l'esercizio, non avevamo molto da eccepire, se non la necessità di fare chiarezza sui motivi che hanno indotto il Governo a disporre la proroga sino alla data del 1° luglio 2009, considerato che la gara per l'assegnazione della nuova concessione si è conclusa nel mese di febbraio di quest'anno e da quel momento decorreva il termine di sette mesi per l'attuazione degli impegni dell'aggiudicatario, termine che comunque viene ora dilatato a ben sedici mesi. Ma è sul resto dell'impianto che vogliamo sottolineare alcune nostre preoccupazioni e mi soffermo in particolare su due considerazioni. Una delle finalità contenute nell'articolo 1-*bis* sta nell'obiettivo di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, che imputava al nostro Paese la violazione del principio di trasparenza, avendo rinnovato le 329 vecchie concessioni dell'UNIRE per la gestione delle scommesse ippiche senza aver esperito la gara d'appalto. Ora si introduce una procedura selettiva e si stabilisce che le concessioni siano aggiudicate alle offerte che risultino economicamente più elevate rispetto ad una base minima di 85.000 euro e che invece per i soggetti già titolari di concessione l'importo sia ridotto del 25 per cento con riferimento a quanto indicato nell'offerta. E così rischiamo una soluzione paradossale: ad una sentenza che ci chiede di osservare il divieto di discriminazione e di applicare il principio di trasparenza, si risponde con un provvedimento che - cito testualmente dalla nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato «potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti ammessi alla partecipazione alla gara (...) che potrebbe determinare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria». Capite, colleghi? Nell'uscire da una sentenza si rischia di entrare in una procedura di infrazione. Un capolavoro di coerenza. Credo che il Governo debba fornire chiarimenti precisi su questo aspetto. L'altra motivazione addotta per l'inserimento dell'articolo 1-*bis* sulle scommesse ippiche è quella di dare risposte immediate al settore dell'ippica. Siamo ben consapevoli dell'importanza di occuparsi di questo comparto, oggi entrato in sofferenza, che merita certamente attenzione, parte di una filiera produttiva che interessa migliaia di operatori, di allevatori, che presenta interconnessioni con il mondo agricolo, zootecnico, industriale, sportivo, con il settore della genetica, patrimonio di prestigio e di tradizione per il nostro Paese, eppure, la risposta a queste finalità non mi pare così chiara ed evidente. Oltre ad un contributo di 25 milioni di euro all'UNIRE (ma con quali obiettivi? Quale rigore, quale chiarezza, quale progetto di riforma e ristutturazione dell'ente?), il decreto prevede infatti l'istituzione di un fondo destinato - in modo assolutamente indefinito ed approssimativo all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero alle esigenze finanziarie del CONI e dell'UNIRE ed al bilancio dello Stato per la parte non destinata alle altre esigenze. Diverse finalizzazioni di spesa, quindi, senza tuttavia indicare proporzioni o limiti quantitativi e senza affrontare il vero nodo che è la diminuzione dei redditi di chi opera nel comparto. E nella vaghezza è insito il rischio di non dare risposte adeguate se non solo quelle di bandiera, se non quelle di strizzare l'occhio a qualche interesse particolare. Per tutti questi motivi, siamo convinti che l'urgenza vera sia nella ripresa della ricerca di un ampio confronto di merito e di interventi organici su temi, come abbiamo visto, di portata molto ampia proprio per le implicazioni di ordine etico morale che intersecano l'attività pubblica nel settore del gioco. Su questo siamo pronti come Partito Democratico a fare la nostra parte, a condizione che il Governo a perseguire la strada dell'assenza totale di confronto e di dialogo nelle aule parlamentari dove ormai si consumano frettolosi percorsi di ratifica di decisioni già assunte.

*(IdV)*. Signora Presidente, il decreto oggi in discussione originariamente disciplinava la proroga della concessione per la gestione dell'esercizio dell'Enalotto, dettata dall'impossibilità di aggiudicare nei tempi inizialmente previsti la nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Nel nome del pubblico interesse l'attuale gestore, SISAL, continuerà a garantire la continuità della gestione corrente fino a quando la nuova gestione non entrerà in pieno funzionamento. Ricordiamo che al momento la nuova concessione è in corso di affidamento. A causa dell'unico *hobby* del Governo, cioè quello di utilizzare il decreto‑legge come strumento per macinare nel minore tempo possibile prodotti legislativi, il cuore originario del decreto è stato arricchito da ulteriori disposizioni in materia di giochi di azzardo. Gli emendamenti apportati alla Camera riguardano l'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse di cavalli e gli apparecchi per il gioco lecito, meglio conosciuti come *videopoker* e *slot machine* elettroniche.

mancava però di disciplinare un gioco d'azzardo che negli ultimi anni si è rapidamente diffuso nella società italiana fino a diventare oggi un fenomeno di tale portata da non poter essere tralasciato nella riorganizzazione di materie definite come urgenti per il loro impatto diretto sulla società.

Il gioco a cui mi riferisco, onorevoli colleghi, è quello del bingo: un gioco praticato su tutto il territorio nazionale e che richiede l'immediata definizione di parametri di regolamentazione più precisi per la tutela del cittadino, soprattutto in un momento storico in cui la crisi economica ci sta portando a vivere situazioni di estrema vulnerabilità che si riflettono direttamente su una maggiore precarietà degli assetti sociali. Proprio questo emendamento mi risulta

Il bingo è in ogni caso un gioco d'azzardo a tutti gli effetti che, come gli altri giochi d'azzardo suoi cugini (spaziando dalla cinematografica *roulette* al più prosaico *videopoker*) possono trasformarsi da abitudine in vizio. Il vizio, a sua volta, può degenerare e portare a dipendenza e disturbi patologici, con pesanti conseguenze sulla condizione economica di coloro che iniziano a soffrire di questa patologia di gioco. La dipendenza patologica dal gioco d'azzardo è un fenomeno molto sottostimato in Italia - e ahimè anche da questo da questo Governo, voglio sottolinearlo - che affligge addirittura il 5 per cento circa della popolazione, ovvero 30.000 italiani, sviluppando una dipendenza psicofisiologica, simile a quella indotta da sostanze stupefacenti.

a dire la fascia di popolazione notoriamente più debole dal punto di vista economico. Tutti questi elementi, legati al gioco d'azzardo, assumono tonalità ancora più cupe se vengono considerati alla luce dell'attuale momento di crisi che il nostro Paese sta attraversando. Infatti, soprattutto nei momenti di crisi che la mancanza di prospettive porta molte persone - ahimè! - a rifugiarsi nel gioco, riponendo nella «dea bendata» l'ultima speranza di risollevare la propria situazione. É questo che dobbiamo bloccare e dovrebbe appunto essere questa la responsabilità di un Governo. La patologia del gioco in questa situazione un terreno molto fertile per degenerare e creare fenomeni di deriva sociale di intere famiglie ridotte al lastrico: e per fortuna che questo Governo aiuta le famiglie! Qui si tratta, invece,

quella speranza che lega tante famiglie nel modificare il proprio futuro affidandosi al gioco. Vorrei ricordare, signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, che soprattutto nei momenti di grave crisi economica, come l'attuale, sempre più famiglie di lavoratori, pensionati

dalla propaganda di quella cattiva maestra della TV pubblica che dispensa pacchi serali nei programmi più ascoltati, invece di proporre cultura. Quindi, milioni di cittadini, soprattutto dei ceti meno abbienti, affidano la loro speranza alle tante scommesse, dal superenalotto, alle schedine, ai giochi nuovi, nell'illusione di risolvere i duri problemi quotidiani. In tale contesto, il Governo, con il decreto‑legge n. 149 del 2008, Atto Senato n. 1196, anziché disciplinare alcuni fenomeni di dipendenza dal gioco

fanno notizia, alimenta le scommesse teorizzando e rafforzando il concetto di Stato biscazziere.

nell'ennesimo decreto «la previsione - quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva - di una scadenza della concessione successiva al 31 gennaio 2009 sembrerebbe finalizzata a precludere la partecipazione di quei soggetti titolari di concessioni la cui proroga è stata giudicata illegittima dalla Corte di giustizia CE e, di conseguenza, revocate a decorrere dal 31 gennaio 2009. È presumibile che i titolari di concessione con scadenza successiva al 31 gennaio 2009 siano in possesso di idonei requisiti di affidabilità già accertati al momento di affidamento delle medesime concessioni». Noi, quindi, e mi avvio alla conclusione signora Presidente, diamo un giudizio molto severo su questo provvedimento perché

richiama, dicendo che si è persa l'ennesima occasione per dialogare con l'opposizione democratica.

dalla quale è consentito il gioco del Lotto, dell'Enalotto e del Superenalotto. Sappiamo comunque, come ha detto il Governo in Commissione, che esiste un impegno preciso ad intervenire e disciplinare la materia con una

mi permetto di dire che al collega Pedica che mente e che sa di mentire quando dichiara che in Commissione è stato bocciato l'emendamento sul bingo. emendamento, carissimo collega, è stato ritenuto inammissibile perché non confacente con la materia oggetto del decreto. Allora bisogna essere sinceri con noi stessi e con chi ci ascolta, se vogliamo fare un servizio

stata uno scivolone - mi auguro - per una cattiva informazione o perché non abbia voluto adeguatamente informarsi; non voglio pensare il contrario perché sarebbe particolarmente grave. *(Applausi

un *incipit* legato a due punti che hanno caratterizzato - e devo dire personalmente pensavo in modo positivo - l'avvio dell'attività del Governo. Mi riferisco alla semplificazione normativa, e quindi all'aver addirittura individuato un Ministro *ad hoc*, e all'efficientamento della pubblica amministrazione. Due temi che trovano indiscutibilmente d'accordo maggioranza e minoranza nel ritenerli fondamentali per migliorare profondamente la qualità della nostra normazione e dell'organizzazione del nostro Paese.

che non più di un ventesimo del contenuto di questa norma è riferito alle disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. Quindi credo che questa sia una vera norma pullman, vale a dire un titolo all'interno del quale è stato poi inserito tutto ciò che di volta in volta alle varie fermate, per svariate esigenze molto lontane dal titolo stesso, si verificava e quindi si rendeva opportuno aggiungere. Questa non è semplificazione normativa. Allora, se la semplificazione normativa, su cui abbiamo fatto grandi proclami, si concretizza nel fatto che si semplifica il passato e si complica il presente per perpetuare la specie, devo dire che è vero che abbiamo innovato ma con la semplificazione normativa a tela di Penelope: semplificare il passato e procurarci materiale per il futuro non è esattamente quello che noi si intendeva nel dire che è buona cosa avere un programma di semplificazione normativa. Vengo all'efficienza, che è il secondo aspetto. Il punto prima reca, con grande evidenza, il nocciolo della problematica che trattiamo, ossia la proroga. Con il provvedimento in esame si concede una proroga alla SISAL S.p.A per la gestione di una serie di attività. proroga non è mai sinonimo di efficienza; una proroga può essereconcessa una volta perché si verificano delle condizioni contingenti che la rendono necessaria. Siamo alla quinta

gli atti di cui oggi parliamo per altro tempo. La Relazione tecnica prevede che il nuovo concessionario non può essere ancora nella pienezza della sua attribuzione perché deve sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari atte a garantire l'idoneità della nuova organizzazione, nonché la loro conformità a progetti presentati in gara. che si è presentato un soggetto che ha vinto la gara - erano tre i soggetti che si presentavano - il quale deve verificare se poi è in grado di fare ciò per cui ha vinto la gara Credo che neppure nell'assegnazione delle matite in una normale pubblica amministrazione si accetterebbe che il fornitore individuato dimostri in seguito di essere in grado di fare non non una banale fornitura di matite, ma una cosa molto più complessa come questa, soltanto dopo aver avuto la gara assegnata. Quindi, in questo caso, abbiamo una proroga che va addirittura fino al luglio del prossimo anno e ci rivedremo a luglio del prossimo anno per capire cosa è successo e quali costi saranno conseguenti al non aver assicurato prima un adempimento

sicuramente ci sarà anche il problema di un ulteriore costo che la norma ingenera rispetto ad un contenzioso da complicazione normativa. Ebbene, è il contenzioso che si innesca nel momento in cui si prevede che, qualora i soggetti aggiudicatari della gara aperta per 3.000 concessioni

questo - si può già dire oggi - è in aperta violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza. È palese che su questo si aprirà un contenzioso che complicherà, ritarderà e costerà per le sanzioni che subiremo. Questo lo diciamo oggi

L'articolo aggiuntivo 1-*bis*, al comma 7, istituisce un fondo che è alimentato dalle maggiori entrate determinate dalla raccolta e che è destinato alle esigenze finanziarie relative alle attività istitutive di CONI e di UNIRE. Ed aggiunge che a quest'ultimo è assegnato per l'anno 2008 un contributo pari a 25 milioni di euro.

Credo che in una normale gestione, da quella familiare a quella aziendale, prima di conferire nuove risorse si chiede conto dell'utilizzo di quelle esistenti. non molti anni fa con una norma del 2003 è stato concesso un mutuo di 150 milioni di euro all'UNIRE dalla Cassa depositi e prestiti con oneri a parziale carico dello Stato. credo che prima di passare all'assegnazione di ulteriori risorse per le stesse finalità, poteva rendersi del tutto opportuno una *due diligence* normale per capire quale fossero i risultati di quell'impegno di risorse pubbliche e quindi quali fossero le ragioni che rendono oggi necessario questo ulteriore intervento con questa somma. L'ultima cosa su cui richiamo la vostra attenzione, signora Presidente, è questa: 25 milioni di euro in tempi di casse molto magre e quindi di grandi difficoltà a reperire risorse dove vengono reperiti? Vengono reperiti su un fondo destinato all'estinzione di debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato. Ricordo, al riguardo, soltanto che certamente il fondo non conterrà quanto sufficiente a risolvere il problema, ma le amministrazioni pubbliche

Il decreto-legge al nostro esame reca disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, ma prevedeva, nel suo testo originario, un'unica disposizione in tema di esercizio del gioco Enalotto. La gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha condotto all'individuazione di un nuovo concessionario (SISAL S.p.A.) che, tuttavia, non può essere ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, perché si deve attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari che garantiscano l'idoneità della nuova organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara. Dunque, considerata la scadenza del termine della concessione del gioco Enalotto (30 settembre 2008), si è resa obbligatoria l'adozione di una proroga utilizzando un provvedimento avente forza di legge, affinché non venissero meno per il concessionario i titoli abilitativi all'esercizio della raccolta, con danni irrecuperabili in termini di mancate entrate erariali e di perdita di avviamento del gioco stesso. Pertanto, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, conseguentemente all'approvazione di due emendamenti governativi, a loro volta modificati attraverso l'approvazione di subemendamenti. 1-*bis* interviene nel settore delle scommesse ippiche e sportive, autorizzando l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a realizzare un'apposita procedura selettiva, aperta ai soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea, per la concessione, fino al 30 giugno 2016, del diritto del diritto di esercizio e raccolta, in rete fisica, di giochi su base ippica e sportiva, nel limite massimo di 3.000 soggetti abilitati alla raccolta. L'articolo 1-*ter* rimette ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari - la disciplina relativa alla sperimentazione degli apparecchi elettronici per il gioco lecito collegati in rete.

per il 2009 di 23 miliardi di euro, lo 0,7 per cento ammonta a 161 milioni di euro. La crisi del settore dell'ippica è dovuta principalmente al calo di scommesse. Le corse dei cavalli non appassionano più: dal 2003 ad oggi il totale degli euro raccolti è passato da 2,9 miliardi di euro ai 2,6 miliardi

di raccogliere le giocate passando dai vecchi bar dove si giocava la schedina o dalle vecchie ricevitorie a sale scommesse più attrezzate, ma l'unico risultato ottenuto è stato quello di far passare da 20.000 a 6.000 i punti vendita per le scommesse. Si è reso, dunque, necessario un intervento che garantisse attenzione per un settore in crisi nel quale operano circa 50.000 addetti: non solo fantini ed allevatori, ma tutta la filiera interessata.

Vero è che il provvedimento viene ad incidere su un comparto di gioco. Bisogna certamente prestare attenzione anche al settore degli apparecchi che dal 2004 si sta gradualmente riprendendo a seguito della bonifica del territorio dalla presenza dell'illegalità diffusa dei vecchi *videopoker* e della malavita organizzata. Quindi il provvedimento, cosi come modificato cosi come modificato dalla Camera dei deputati, mira a salvare un comparto in crisi. Ovviamente bisogna evitare di generare altra crisi, che rischia di risultare irreversibile. La soluzione per il salvataggio dell'ippica è un punto di equilibrio. Certo è importante ribadire che non deve passare il principio per cui un settore specifico possa finanziare un altro in crisi. Con questo obiettivo, il sottosegretario Gìorgetti ha già annunciato un imminente disegno di legge, di iniziativa governativa, volto a disciplinare le possibilità di effettuare scommesse e giocate *on line.* Si tratta di un comparto che certamente necessita di una normativa quadro a livello nazionale che, mettendo il settore in sicurezza, può renderlo una grande opportunità. Sarebbe quindi auspicabile che tale iniziativa potesse costituire l'occasione per omogeneizzare e armonizzare il prelievo tributario su tutte le forme di gioco, con particolare attenzione all'equilibrio tra i vari comparti, e contemperando le esigenze di gettito con quelle di rilancio dell'intero settore. Il ministro Zaia ha anticipato l'istituzione di una commissione di lavoro con i rappresentanti del settore.

escano dall'ambiguità e si decidano, una volta per tutte, a misurarsi con il nostro mercato alle stesse condizioni con le quali operano tutti i soggetti concessionari. Il tutto nel rispetto di quella linea annunciata dal Governo

colleghi, chi come me ha sufficiente milizia di partecipazione a questa Assemblea ha avuto la possibilità nel tempo di vedere germogliare e dilatare il fenomeno dei giochi di Stato, non sempre condiviso, spesso contrastato, anche per motivi di ordine ideologico e religioso, ma alla fine accettato in funzione di un processo di globalizzazione che aveva investito il settore e che, se non fosse stato adottato e disciplinato anche in Italia, sarebbe stato subìto per la via Internet. È per questo motivo che il nostro Paese ha dovuto e ha voluto alla fine accettare e regolamentare questo importante settore, che determina un comparto notevole delle entrate dello Stato. Per questo provvedimento ringrazio il Governo e più segnatamente il relatore, che ci ha dato in Commissione una corposa relazione e ci ha aiutato a comprendere quanto segue.

ben 329 agenzie ippiche che raccoglievano scommesse di gioco. Per questa via, noi avremmo dovuto o potuto provvedere sin dal 2006. Siamo al 2008; evidentemente un po' di tempo se l'è preso il Governo precedente, un po' meno questo Governo, vero che entro la fine dell'anno, così come ha anticipato il rappresentante del Governo, sottosegretario Giorgetti, avremo un disegno di legge che riordinerà tutta quanta la materia. Quindi, facciamo presto perché è necessario mettere ordine, come d'altra parte sin dal 2007 aveva detto la sentenza della Corte di giustizia. L'armonizzazione per poter consentire la sportività con il gioco propriamente detto nel comparto ippico pure si appalesa necessaria per questo settore, che al momento può non riguardare me,

appassionati, non perché giochiamo ma perché ormai questa entrata dello Stato è così notevole e cospicua che merita tutto il nostro e il vostro rispetto.

colleghi, udito il parere della Giunta per il Regolamento, reso all'unanimità nella riunione di questa mattina, la Presidenza ha proceduto all'integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento. Sono stati pertanto chiamati a far parte della Giunta per il Regolamento i senatori Felice Belisario, Gianpiero D'Alia, Giovanni Pistorio e Paolo Tancredi. finestra"). Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.